della sospensione degli sfratti fino al 15 ottobre, secondo i criteri sociali e territoriali definiti dalla legge n. 9 del 2007, impostata proprio in quest'Aula; in secondo luogo, perché il provvedimento alcune norme sul terreno dei diritti previdenziali, della tutela dei lavoratori contro i licenziamenti individuali e, più in generale, in materia di ammortizzatori sociali. A questi aspetti si aggiungono alcuni altri elementi positivi, già elencati stamattina dal collega Albonetti, a partire dalla

mancata, evidenziata dal senatore Salvi nel suo intervento sull'ordine del giorno relativo al problema dei salari, in quanto sarebbe stata possibile la piena attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della finanziaria per aumentare il salario reale dei lavoratori

altro che passare dalle parole ai fatti! Ad esempio, ci ha stupiti l'atteggiamento del Partito Democratico che alla Camera ha presentato un emendamento, a nostro avviso, non coerente con la lettera e lo spirito della finanziaria 2008. È un emendamento che spalmava la riduzione fiscale su tutti i redditi, non solo su quelli da lavoro dipendente legati ai salari più bassi. È necessario a questo punto, e mi rivolgo al sottosegretario Lettieri che ha seguito i lavori, che nelle

nell'applicazione di quanto previsto dalla legge e rafforzato dall'ordine del giorno approvato dal Senato, anche perché per due anni, nella maggioranza che finora ha sostenuto il Governo, abbiamo affermato che al risanamento andava affiancata la redistribuzione del reddito. Peraltro, sappiamo tutti che il Governo è stato fatto cadere proprio in quest'Aula da forze moderate della coalizione proprio dopo l'approvazione della legge finanziaria, forse per impedire che

(impegno positivo raggiunto da questo Governo) per aumentare il salario reale dei lavoratori, per dare un respiro ai redditi più bassi, e non per prevedere altri fondi a favore delle imprese e altri regali alla Confindustria.

segnalare prevalentemente un problema di metodo, cioè la necessità di legare sempre manovre che incidono pesantemente sul bilancio a una verifica complessiva non solo sul saldo netto

quale funzione si scorpora da Sviluppo Italia. A questo proposito ribadiamo quanto previsto dal piano di riordino e dismissione, su cui aveva lavorato molto il collega Villone nella finanziaria 2007;

riconosciuta dalla legge n. 266 del 1991, schiacciando in questo modo il volontariato, che garantisce tanti servizi ai deboli, rispetto a un'organizzazione che ha ben altra ragion d'essere, ben altra finalità e ben altra struttura.

Ebbene, noi desideriamo evitare che migliaia di famiglie siano sfrattate dalle loro case in questi mesi, dando tempo al futuro Parlamento e al futuro Governo di portare avanti il piano per l'edilizia residenziale pubblica, già finanziato e concordato con le Regioni, che dovrà rendere disponibile ogni anno, per dieci anni, 8.000 alloggi, valorizzando quella politica complessiva per la casa a favore dei ceti più deboli che ha rappresentato uno dei punti su cui a nostro avviso l'azione del Governo si è dispiegata con maggior efficacia sociale.

anche perché taroccata da una pessima legge elettorale, che non ha garantito alcuna governabilità. In questo clima di contagiosa irresponsabilità, ognuno - sottolineo, ognuno - ha abdicato ai propri doveri. Questa legislatura e questa classe politica, cari colleghi, verranno ricordate così come fotografate nel *best seller* «La Casta» di Rizzo e Stella, ed il perché è sotto gli occhi di tutti. Anche il desolante squallore di quest'Aula che si appresta a compiere l'ultimo atto di una sfortunata legislatura è un emblema che rende plasticamente l'idea di quanto voglio rappresentare. Ognuno continua a bivaccare in Aula e a interessarsi di altre cose; nel frattempo, signor Presidente, nel disinteresse generale - e a volte, mi consenta di dirlo, anche della Presidenza - si approvano normative che lasceranno un segno tra la gente. Ancora una volta, infatti, il Parlamento sta per licenziare una normativa (queste mille proroghe, che ho ribattezzato le «mille marchette») che è l'epilogo emblematico di un modo indecente di legiferare: nessun interesse reale per il corpo elettorale; nessun rispetto delle regole democratiche che dovrebbero costituire l'alveo di garanzia nel quale ogni istituzione esercita correttamente la propria funzione; nessun pudore nel mettere in campo l'ennesimo assalto alla diligenza della cosa pubblica. Ecco perché, signor Presidente, il provvedimento che quest'Aula si accinge ad approvare

(dalla riapertura dei termini per il finanziamento pubblico ai partiti, fino alla spartizione delle nomine ed alla creazione di inutili, nuove postazioni che serviranno ancor più a determinare uno sperpero ignobile delle pubbliche risorse). È ancor più grave, signor Presidente, che ciò accada nel colpevole ed acquiescente silenzio generale, mentre il nostro Paese soffre per una condizione economica sempre più disastrosa. Ecco perché, quale estremo, disperato atto, avendo verificato ‑ cosa che sto facendo ancora adesso ‑ nel disinteresse generale l'inutilità di ogni richiamo ad un senso di responsabilità ormai scomparso in quest'Aula, mi sono rivolto direttamente al Presidente della Repubblica, per chiedergli, con il rispetto che gli è dovuto, un puntuale esercizio delle sue prerogative. Questo provvedimento (che sconta complessivamente il parere contrario di una Commissione bilancio che è sempre stata filogovernativa, e molto spesso ha coperto pure ciò che non poteva essere coperto) non ha un'effettiva copertura, ed è infarcito di macroscopiche illegittimità di rango costituzionale: non merita, pertanto, di essere promulgato. Le indecenze possono essere coltivate in quest'Aula, ma qualcuno dovrà farsene carico prima che diventino effettive. Non riesco a rassegnarmi, signor Presidente, all'idea di un Quirinale che decide di intervenire quando, con il decreto‑legge sull'*election day*, si toccano le prerogative dei vari partiti, e possa invece rimanere silente quando tutti i partiti insieme ledono inesorabilmente gli interessi del corpo elettorale e le regole sancite dalla nostra Costituzione. Sono convinto che la nostra democrazia e le nostre istituzioni abbiano al loro interno ancora gli anticorpi sufficienti. Non mi rassegno ad un'Italia così e combatterò con tutte le mie forze per cambiarla.

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, questo decreto-legge rappresenta un pessimo atto finale della legislatura. Immaginato come strumento di allargamento del consenso, ha finito per dilatarsi a dismisura. Siete riusciti perfino a innovare le procedure di bilancio, introducendo la terza finanziaria, anziché procedere nel senso dell'autoregolamentazione. Questa, infatti, possiamo considerarla appunto la finanziaria-*ter*, di ben 105 articoli. Non vi sono soltanto proroghe di termini o misure urgenti e necessarie, ma anche norme ordinamentali, come quelle che riguardano la durata dell'*Authority* e quelle in materia di responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche. E qui il pensiero va anche al controllo delle municipalizzate e al cosiddetto capitalismo regionale. Non c'è attenzione al serio problema della *govern**ance* e al regime del doppio controllo, che deriva dal codice civile e dall'azione della Corte dei conti. rileva l'introduzione di scelte discutibili di stampo localistico e assistenziali, cresciute a dismisura. Queste vanno dagli interventi finanziari a quello specifico destinato agli ammortizzatori sociali per le crisi occupazionali - che non risolverà certo il problema di Malpensa, ma ha condizionato l'azione del Gruppo della Lega fino al voto determinante che ha salvato il provvedimento dal possibile ritorno alla Camera alle misure per l'emergenza rifiuti in Campania, agli interventi più consistenti per il Policlinico di Roma (250 milioni di euro sfuggiti all'attento senatore Gramazio). Sull'emergenza abitativa non si è guardato alla realtà ma alla demagogia. Certo, non mancano misure come il credito d'imposta sugli investimenti o quella da noi sostenuta sulla rottamazione auto, che ha superato i veti e l'ostruzionismo dei Verdi. È stata persa però l'occasione per reintrodurre gli incentivi CIP 6 per i termovalorizzatori di tutte le Regioni e non quelli della sola Campania. Condividiamo alcune scelte relative all'edilizia per le Forze armate e alla possibilità per la Croce Rossa di essere riconosciuta nel registro del volontariato, perché consente di dispiegare la vasta azione del volontariato in ambito locale nei limiti della sua specifica attività. È vero che è un provvedimento del Governo modificato pesantemente in sede parlamentare alla Camera. Ciò ha fatto perdere di vista ogni equilibrio finanziario. Sono stati asciugati i fondi globali ipotecando le scelte future. Questo decreto può essere considerato uno sportello elettorale cui molti hanno attinto e che ha determinato non solo il parere formale contrario della Commissione bilancio, ma un effetto pesantemente negativo sul fabbisogno e sull'indebitamento della pubblica amministrazione per il 2008. La mancanza dei prospetti di copertura e adeguate valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, costretta a imbarazzati silenzi, ne sono una chiara dimostrazione. E che dire della sanatoria retroattiva camuffata da deroga per la posizione dei concessionari? Non si sta dalla parte dei contribuenti, ma si preferisce sanare gli errori dei concessionari in violazione dello Statuto del contribuente. Ma l'aspetto più negativo di questo decreto è rappresentato dalla votazione dell'ordine del giorno sull'uso del cosiddetto tesoretto attraverso un decreto-legge per intervenire nel corso della campagna elettorale, come ha sostenuto poco fa l'onorevole Bertinotti, condizionando l'orientamento degli elettori. In quella votazione abbiamo registrato anche il tentativo di continuare nella dilapidazione delle risorse pubbliche prima di una corretta e attenta valutazione del quadro di finanza pubblica, già pesantemente pregiudicato da quelle norme che vi accingete ad approvare, prive di copertura finanziaria. E come sottovalutare il clamoroso errore politico registrato stamani allorquando due partiti, dispiegati nella esaltazione del partito unico, hanno assunto un atteggiamento di voto divergente e contrastante, determinando una crepa pericolosa su comportamenti che avrebbero dovuto avere ben altra linearità e condivisione su scelte fondamentali nella prospettiva dell'azione di Governo che rischia di essere pesantemente condizionata dal voto odierno? È tempo di guardare alla famiglia con misure serie, incisive, profonde, di programma e non estemporanee, alla famiglia come entità fiscale, prevedendo una *no tax area* legata ai bisogni. I partiti non si costruiscono con operazioni di *marketing* elettorale. E allora oggi avrebbe dovuto prevalere rigore e senso di responsabilità in chi ha a cuore il risanamento finanziario del Paese, senza pregiudicare le possibilità di ripresa, un vero autentico comportamento *bipartisan* che prendesse le distanze dalle scelte che vi accingete ad approvare, determinando le condizioni per la decadenza del decreto. Hanno prevalso, invece, i reciproci condizionamenti in analogia a quanto sta avvenendo nei comportamenti elettorali, scaricando gli oneri sulla finanza pubblica laddove la spartizione del contenuto del bottino di questo decreto rappresenta la prova che non hanno prevalso le ragioni del Paese e quelle del bene comune ma la logica degli interessi e delle convenienze. il decreto-legge in esame è il fallimento dell'azione di questo Governo, incapace di affrontare i problemi del Paese, capace solo di dilapidare due anni di crescita, di sperperare un extragettito e di determinare un'inflazione *record* insieme a una pressione fiscale che supera il 44 per cento. Per queste ragioni il Gruppo UDC esprime il voto contrario sul provvedimento, che non affronta i problemi reali del Paese e dimostra l'inefficienza del Governo e della maggioranza.

Signor Presidente, signori senatori, il Gruppo Forza Italia voterà contro il provvedimento in esame che segna il coerente epilogo di una brutta legislatura e di un programma di Governo più impegnato a distribuire prebende che a badare agli interessi degli italiani. L'ennesima brutta pagina di questo Governo. Il decreto è viziato da una insopportabile disomogeneità: tratta di sanità, infrastrutture, immondizie, ricerca, università, materie che avrebbero richiesto tempi di approfondimento e previsioni di bilancio. Ed invece si è inserito di tutto di più, perché agli originari già troppi 51 articoli nel passaggio alla Camera se ne sono aggiunti altri 50 in una sorta di assalto da fine corsa, di assalto alla diligenza e, si badi, senza la presentazione di alcuna scheda tecnica che, ove ci fosse stata, avrebbe fatto emergere seri elementi di criticità finanziaria. Quello che francamente sconcerta, però, è che nella campagna elettorale, che è già iniziata, sentiamo ripetere in maniera monotona, quasi ossessiva, dalla ex maggioranza che è necessario comprimere le spese, che sulle spese ci deve essere il massimo rigore e poi queste restano soltanto parole, inattendibili promesse, il libro dei sogni. I fatti dicono invece il contrario. Le uscite extra di questo decreto sono valutate in circa 1 miliardo di euro; in larga parte sono senza copertura finanziaria. Ciò significa che tutte queste spese peseranno poi sulle tasche degli italiani. un disastro contabile che si aggiunge al quadro economico desolante lasciato dal centro-sinistra, un tasso di crescita per il 2008 pari allo 0,7 un tasso di inflazione pari al 2,9 per cento, un *deficit* PIL pari al 2,7 per cento e un livello di pressione fiscale - il livello massimo toccato negli ultimi anni - pari al 44 È il quadro di una Italia in ginocchio, definita di recente - non certamente da noi - maglia nera in Europa. È il quadro di una Italia dove il centro-sinistra ha aumentato rovinosamente i livelli di povertà. Noi voteremo contro questo provvedimento che danneggia pesantemente l'economia senza produrre alcun beneficio, senza elargire alcun servizio agli italiani.

Non siamo stati paralizzati. Come opposizione non abbiamo paralizzato questo ramo del Parlamento, anche se avremmo potuto farlo ricorrendo all'ostruzionismo. Ci siamo fatti carico di svolgere un ruolo d'opposizione responsabile

Questa legislatura resterà - credo - indimenticabile nella storia del nostro Paese, sia per la sua brevità - penso si tratti della legislatura più breve della storia - sia per lo scenario numerico, che ha visto contrapposte due coalizioni che si sono misurate sul filo del rasoio. Vi è stata poi l'anomalia dell'essenzialità del voto dei senatori a vita, che ha costituito anche motivo di dibattito politico. Mi auguro che il tema da noi evidenziato dell'essenzialità del voto dei senatori a vita,

e in grado di trovare la soluzione ai veri nodi strutturali che necessitano di un miglioramento e di un ammodernamento delle nostre istituzioni. Con questo mio auspicio le rinnoviamo

augurandoci che la campagna elettorale abbia toni contenuti e non sia aspra, una campagna elettorale corretta che si misuri sui progetti, sui programmi e non sulle offese personali.

del Parlamento, come alla Camera dei deputati, siamo stati eletti secondo uno schieramento di scontro tra alleanze elettorali. La prossima legislatura sarà caratterizzata da una straordinaria novità: in Parlamento non ci si presenterà più come portatori di due schieramenti alternativi elettorali, ma come portatori di esigenze politiche distinte le une dalle altre. Da questo punto di vista, la vostra esperienza sarà molto importante, la riterrei conclusiva di un'esperienza terminata, quella di un sistema elettorale nel quale ci si è scontrati dal 1994 in poi, e di apertura di una nuova stagione nella quale ci si confronterà

approvato un decreto sulla sicurezza. Allora, o lo lasciamo decadere oppure ci ritroveremo ancora una volta qui a lavorare. In ogni caso, mi associo a quanto dichiarato dal presidente Schifani.

se potessimo, come tante altre cose della legislatura, ma questa in particolare. Purtroppo non sarà possibile, perché ce lo ricorderà la tragica realtà dei conti pubblici. un provvedimento di 4 miliardi di euro, che avete lanciato come possibile ciambella di salvataggio per evitare il naufragio

un comma introduce un contributo per quelle orchestre, o quant'altro, che in qualche modo si trovassero in difficoltà. Non si sa a chi andrà, non si sa di quanto sarà l'importo, ma sarà tanto. abbiamo la campagna elettorale di quello che prima era candidato, perché ve li scambiate, la campagna elettorale di Roma. Cosa c'è di meglio che dare bazzecole, ovviamente - 250 milioni di euro al Policlinico Umberto I? È una cosa che grida vendetta e di cui

della Padania sana che non ha bisogno di vivere a carico dello Stato, che chiede di poter vivere in pace del proprio lavoro, di essere lasciata in pace da questo Stato parassita, che chiede fortemente che il Governo Prodi e quello del suo accolito Veltroni se ne vada e tolga il disturbo. *(Applausi Alleanza Nazionale con i suoi senatori nelle Commissioni ed in Aula ha agito con molta correttezza e soprattutto con responsabilità perché, se è vero che in questo provvedimento ci sono punti che potevano essere assegnati alla normale procedura legislativa, vi è anche da dire che vi sono problemi urgenti e necessari cui il Governo e questo Parlamento stanno dando risposte urgenti.

Questo non significa che diamo un parere positivo al provvedimento di per sé. Si tratta di un modello di produzione normativa su cui altre volte abbiamo avanzato critiche da tutte le parti, ma certamente non ci possiamo limitare a fare le verginelle offese per iniziative alle quali abbiamo contribuito anche noi negli anni passati o comunque anche in questa legislatura che volge al termine. Dico che facendo le verginelle offese offese non si risolve il problema. Siamo pronti a metterci attorno ad un tavolo, a vedere le modalità che giustificano l'urgenza e la necessità, trovando uno strumento di immediata risposta ma che sia legittimo nelle procedure e sentito dalla gente. gente. È vero che con questo provvedimento si risolvono problemi importanti, ma altri significativi non hanno trovato risposta. Mi rendo conto che non basta l'ordine del giorno, anche se accettato

norme utili e necessarie in vista della chiusura anticipata della legislatura e anche se qualche punto ha sollevato talune problematicità credo

il lavoro faticoso di questi mesi, che sono stati importanti anche per il modo con il quale il Senato ha saputo fronteggiare, sia pure in una condizione che potremmo definire costantemente emergenziale, gli impegni che il lavoro del Governo e l'elaborazione delle stesse Aule parlamentari hanno imposto di affrontare. Desidero poi ringraziare gli uffici, per il contributo prezioso e competente che hanno prestato ai Gruppi parlamentari. Voglio ringraziare, infine, i colleghi tutti: non solo quelli del mio Gruppo, non solo quelli della maggioranza, ma anche quelli dell'opposizione. Certo, resta un rammarico: un rammarico: se questa legislatura fosse durata ancora qualche mese, il Parlamento che verrà tra poco eletto dagli italiani sarebbe stato in grado di assicurare al Paese e al prossimo Governo una stabilità ed un'efficacia dell'operare non costretta entro i limiti delle maggioranze risicate determinate dal meccanismo elettorale della legge che ancora governerà le prossime elezioni. Ritengo che ciò rappresenti un'occasione mancata, non soltanto per questi senatori o deputati, o deputati, perché rischia di riconsegnare il Paese ad una situazione di fragilità, di instabilità, ad un vivere effimero delle prossime Camere, incalzate peraltro dalla consultazione e dal voto referendario. però, non può esimermi oggi dal salutare i colleghi che con noi hanno lavorato, pur nell'asprezza del conflitto o nel legittimo tentativo di compiere attività di interdizione anche solo con la continua richiesta di verifica del numero legale, come è nel dovere direi di ogni opposizione. Vorrei ringraziarli davvero per il lavoro che abbiamo compiuto ed augurare a tutti loro un'ottima un'ottima campagna elettorale.

intervengo per esprimere il mio punto di vista difforme da quello che è stato manifestato

abbiamo assistito ad un dibattito ipocrita in Senato ed anche nell'altra Camera, perché quando l'opposizione dichiara di essere contraria e di voler votare contro sa bene che questo decreto è figlio

Da questo punto di vista, per favore, evitiamo almeno l'ipocrisia che questo sarebbe l'ultimo atto del Governo e pertanto bisogna votare contro; sono scelte che se non ci fosse stato l'accordo di tutti non si troverebbero all'interno del provvedimento Detto questo, e solo per manifestare tale malessere, dichiaro che voto per puro spirito di appartenenza e solidarietà al Gruppo.

ho fatto inappropriatamente riferimento al suo lodo sulla trasformazione degli ordini del giorno inammissibili, riferendomi ad essi come alla trasformazione in un invito al Governo. Ho ribadito questo riferimento, ma lo intendevo - l'ho detto in quell'occasione e lo ribadisco adesso - soltanto in merito agli emendamenti che venivano trasformati in ordini del giorno e non già agli ordini del giorno nati e votati favorevolmente in quanto tali. Fatta questa precisazione, Presidente, solo per la chiarezza del verbale, voglio ringraziare la presidente Finocchiaro per avermi dato l'incarico di responsabile del Gruppo del Partito Democratico in seno alla 1a Commissione,

Grazie a tutti e buon lavoro.

ringrazio il Segretario generale e tutti i collaboratori. Dico solo una parola: anch'io ritengo che, nelle condizioni date dai cittadini che ci votarono nel 2006, questa Camera, pur con difficoltà, è riuscita, tirando tirando le somme, a fare il proprio dovere, anche se qualche volta proprio tra i nostri componenti - ma conosco la propaganda politica - c'è stato chi ha sostenuto il contrario. Di questo ringrazio tutti e vi rivolgo un caro augurio.

secondo quanto era stato previsto. Grazie a tutti